L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Onorevoli colleghi, prima di dare avvio ai nostri lavori, desidero manifestare la solidarietà di tutto il Senato e mia personale ai familiari, ai colleghi, agli amici di Helen Joanne Cox, parlamentare britannica barbaramente uccisa giovedì scorso. Jo Cox era stata eletta alla Camera dei comuni per il partito laburista nel 2015, rappresentava la circoscrizione del West Yorkshire, dove era nata. Ha esercitato il proprio mandato con coraggio e determinazione. Come ha detto una sua collega di Westminster, considerava il Parlamento come uno strumento per battersi a favore di tutte le persone nel mondo che più hanno bisogno di noi. Jo Cox aveva infatti a cuore la sorte dei più deboli, degli ultimi, i cui problemi aveva conosciuto da vicino collaborando con imponenti e importanti organizzazioni non governative internazionali, quali Oxfam e Save the children. È stata una giovane e determinata portatrice dei valori della democrazia e della solidarietà. Interpretava il suo ruolo di parlamentare come un mezzo per garantire una giustizia sociale vera, sia fuori che all'interno dei confini nazionali. Proprio mentre dialogava con i cittadini su questi temi è stata uccisa in ragione delle sue idee politiche e del suo impegno. La sua morte, per mano di un estremista, ci induce a manifestare la più ferma condanna nei confronti di qualsiasi fenomeno di intolleranza, specie quando sfocia in atti di così drammatica violenza. Jo Cox lascia un marito e due bambini. A loro in particolare rivolgo l'abbraccio di tutta l'Assemblea del Senato e mio personale. Invito ad osservare un minuto di silenzio.

Signor Presidente, anch'io, a nome delle senatrici e dei senatori del Partito Democratico, desidero abbracciare il marito e i figli di Jo Cox, deputata laburista assassinata in Gran Bretagna la settimana scorsa. Le indagini di Scotland Yard ci diranno se ad ucciderla è stato un pazzo, un esaltato o un criminale comune, ma noi sappiamo già con certezza che il suo è stato un delitto politico. È stata vittima di un assassinio politico, Grazie il suo partito laburista, il suo ideale europeo, l'Europa tutta e quindi anche tutti noi che siamo europeisti. Credo - e voglio dirlo al termine di questo brevissimo intervento - che il suo sacrificio debba spingerci ad una politica migliore e farci capire la necessità di bandire dai nostri dibattiti ogni forma di odio, ogni forma di eccesso, ogni conflitto esagerato. ci deve spingere a cercare sempre modi di convivenza politica quanto più possibile civili e sempre rispettosi delle opinioni l'uno dell'altro. Anche così, penso, noi onoreremo il ricordo, la memoria e l'azione politica di Jo Cox.

la volontaria o l'attivista, come si dice in Gran Bretagna. Si era occupata degli immigrati musulmani, per integrarli, si era occupata molto dei bambini dei bambini e anche dei rapporti fra le religioni, la religione cattolica e la religione protestante, che non sempre vanno d'accordo in Gran Bretagna e, nelle comunità, queste divisioni pesano, pesano enormemente. Era, come si dice, una deputata del collegio, il suo West Yorkshire, come lei ha ricordato, signor Presidente. Nel suo collegio tornava spessissimo, continuamente e, quando ritornava, incontrava le persone. Come diceva giustamente il senatore Zanda, bisogna chiedersi cosa l'abbia uccisa. L'ha uccisa la competizione politica? La posizione, peraltro legittima - che io naturalmente non condivido - di chi vuole separare la Gran Bretagna dall'Europa? No, non è questo. L'ha uccisa l'odio, che sta crescendo enormemente in questo momento nel mondo e purtroppo anche in Italia; un odio che nel mondo anglosassone e in quello francese sta crescendo molto di più che in altre parti del mondo occidentale, del nostro mondo molto sviluppato. Grazie

vengono minacciate. E, quando ci si sente minacciati, il rischio dell'odio è molto forte. Perché è stata uccisa Jo Cox? Lo dico semplicemente: innanzitutto, perché era una donna e, nei periodi di crisi, la donna continua ad essere il nemico, l'emblema di qualcosa che ha avuto successo e che io odio, se non sono d'accordo con lei. Non dimentichiamo queste antiche ferite. In secondo luogo, è stata uccisa perché, figlia di un operaio, si era laureata molto bene in una delle migliori scuole inglesi ed aveva avuto successo. In terzo luogo, perché era una donna con le sue idee ed era stata scelta dal collegio del West Yorkshire. Insisto su questo la democrazia britannica è fondata sul rapporto diretto tra il parlamentare e il suo collegio. È Jo Cox che avrebbe portato il premio di maggioranza avrebbe portato il premio di maggioranza al suo *Premier* anche se, in questo caso, non è stato così perché, come sapete, il premio di maggioranza è poi toccato al partito avverso al partito laburista, cioè al partito di Cameron. Ella aveva quindi un forte radicamento nel suo territorio e nel suo collegio ed era riconosciuta dalle persone. L'uomo senza radici, l'uomo emarginato, il suo assassino, l'uomo che si è alimentato su testi razzisti americani e che ha partecipato ad un *club*, o almeno leggeva la rivista di questo Springbok Club, che è una rivista non solo razzista, ma che propone la segregazione razziale, questo tipo di uomo non sopporta che una donna abbia avuto successo, che una donna si sia guadagnata una promozione sociale, che una donna abbia il consenso politico e sociale. Questa è la realtà con cui dobbiamo fare i conti. Il modo migliore di onorare Jo Cox non è ora semplicemente tirare un sospiro di sollievo, perché sembra che i numeri siano cambiati e sembra forse che il pericolo, temutissimo dalle borse e dai mercati, della

che è in corso nel mondo. Queste piaghe antiche sono appunto l'odio e l'estremismo, che può essere di tipo nazista o di tipo islamista, ma che ha spesso delle radici assolutamente analoghe nella nostra terra. terra. Vorrei concludere con una frase che apparentemente non c'entra: Barack Obama ha detto, a proposito di un'altra strage negli Stati Uniti che questo nemico è interno, è di casa nostra. Ebbene, sappiamo che anche il veleno che ha ucciso Jo Cox è di casa nostra.

di Jo Cox e dei colleghi del Parlamento di Londra di fronte a questo omicidio che lascia sgomenti.

rappresenta una rabbia che non porta comunque da nessuna parte. Inoltre, il fatto che si sia scatenata contro un membro del Parlamento più antico Parlamento più antico del mondo, così come lo conosciamo, è significativo dell'importanza Grazie verbali e dialettici sono all'ordine del giorno, ma purtroppo non sono così rari gli esempi di persone che hanno subito ben più di questo, come è accaduto anche in Italia ancora nel Dopoguerra. Pertanto, il pensiero va all'intera nazione del Regno Unito, chiamata in questi giorni a una scelta molto impegnativa, a tutti coloro che si impegnano attivamente nella politica, con sincerità e con grande disponibilità, nella più viva riprovazione di qualunque tipo di violenza o di incitamento alla violenza per ragioni politiche. La morte di questa giovane e attivissima deputata sia di incitamento a tutti coloro che intendono portare avanti con coraggio e determinazione i loro ideali

Signor Presidente, anche io sono stato colpito, come tutti noi del Movimento 5 Stelle, dall'uccisione della deputata inglese Cox, di cui - guarda caso - pochi giorni prima leggevo l'ultimo intervento pubblico, che era una condanna nei confronti del Regno Unito, responsabile, secondo lei, di un traffico d'armi con l'Arabia Saudita quelle armi che vengono utilizzate nella guerra dello Yemen anche contro la popolazione civile e i bambini, della cui denuncia anche noi del Movimento 5 Stelle ci siamo fatti carico. Grazie

purtroppo, da Gandhi a Malcom X, a Martin Luther King, a Rosa Luxemburg a tanti altri, come Olof Palme. Sono tutte persone che si battevano per l'affermazione della pace

Anche la deputata Cox è rimasta vittima dell'ideologia del colpire chi disturba i manovratori

Signor Presidente, anche i senatori del nostro Gruppo si inchinano commossi alla memoria dell'onorevole Cox. Sulle circostanze della sua morte e di questo odioso assassinio non c'è nulla da dire, in quanto tutto sarebbe esageratamente poco o esageratamente troppo. Resta, se non la memoria per chi non ha avuto modo di conoscerla, l'immagine

alla nazione britannica, attesa da un civile e democratico confronto che non meritava questa pagina dolorosa. Siamo però

che è non la società civile nel senso ansiogeno e scomposto del continente, ma qualche cosa che implica,

di partecipare all'atto istitutivo fondamentale di questo importante istituto internazionale di credito. [ROMANI

di un voto cui si può pervenire abbastanza velocemente, così da essere sicuri di poter affrontare le mozioni sugli stabilimenti balneari immediatamente dopo e quindi oggi pomeriggio.

per gli investimenti in infrastrutture. La predetta Banca, che poi indicherò con l'acronimo AIIB, è una nuova istituzione finanziaria, creata il 29 giugno 2015 a Pechino da parte dei delegati di 50 Paesi aderenti, con il compito di promuovere lo sviluppo economico dell'Asia, ancora gravata da profonde carenze infrastrutturali, attraverso investimenti in infrastrutture, in particolare mediante operazioni di sostegno finanziario - prestiti, partecipazioni al capitale e garanzie - nei settori dell'energia, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle infrastrutture rurali e della logistica urbana. Tra gli Stati fondatori, oltre ovviamente a molti Paesi asiatici, ci sono quattordici Paesi dell'Unione europea (tra cui Regno Unito, Francia e Germania), altri Paesi europei come Svizzera, Norvegia e Islanda e poi tre Paesi extraeuropei, particolarmente importanti (Brasile, Egitto e Sud Africa). Non hanno invece aderito alla nuova istituzione, tra gli altri, gli Stati Uniti e il Giappone. Lo Statuto della nuova Banca asiatica prevede una collaborazione con le altre banche di sviluppo multilaterali, soprattutto con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, la Banca europea per gli investimenti e la Banca mondiale. La AIIB, che ha sede a Pechino e sta avviando in questi mesi le proprie attività, avrà inizialmente a disposizione un capitale di circa 100 miliardi di dollari, di cui il 20 per Ai Paesi asiatici è riservata una quota del 75 per cento del capitale. Le quote di partecipazione dei singoli Paesi sono state determinate mediante una formula che fa riferimento al Prodotto interno lordo, all'interno di ciascuna area regionale. Il maggiore azionista è ovviamente la Cina, seguita da India e Russia. L'Italia è il quinto sottoscrittore tra i Paesi non regionali, dopo Germania, Francia, Brasile e Regno Unito. L'Accordo istitutivo, composto da un preambolo, da 60 articoli e da due allegati, disciplina - fra gli altri - scopo e funzioni dell'istituzione (capitolo I), gli aspetti relativi al capitale (capitolo II), alle operazioni (capitolo III), alle finanze (capitolo IV), alla struttura di governo Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di 5 articoli, che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla quota di partecipazione italiana alla Banca, alla copertura finanziaria e all'entrata in vigore. Da segnalare, signor Presidente, soprattutto l'articolo 3, che riguarda la quota di partecipazione del nostro Paese. Tale quota è pari a 2,57 miliardi di dollari, di cui il 20 per cento deve essere versato. Il disegno di legge autorizza poi il Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare le necessarie operazioni per la copertura finanziaria degli oneri previsti. Gli oneri economici per l'Italia sono stimati in complessivi 515 milioni di euro, di cui 206 per l'anno 2016 e 103 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019. Segnalo che, durante l'esame alla Camera dei deputati, sono stati approvati alcuni emendamenti, di natura essenzialmente tecnico-contabile, e alcuni importanti ordini del giorno. Alcuni colleghi avevano infatti paventato il rischio che la partecipazione italiana alla Banca potesse rappresentare una minaccia alla nostra sovranità o una delega in bianco rispetto alle politiche che la Banca adotterà per la selezione dei progetti sui cui investire. Accogliendo tali ordini del giorno, il Governo si è comunque impegnato a vigilare sulla destinazione dei fondi che affluiranno alla Banca, informando in merito, doverosamente, il Parlamento. Nell'ambito della partecipazione alle decisioni sulle principali politiche operative e finanziarie della Banca, il Governo dovrà anche sostenere, ove possibile, il finanziamento di progetti che privilegino l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili e la riduzione dell'impatto antropico, nell'ottica del modello dell'economia circolare. In realtà, l'adesione del nostro Paese all'Istituto potrebbe costituire una scelta strategica importante, anche con riferimento al nuovo quadro finanziario globale, segnato dal moltiplicarsi dei soggetti e dallo stesso superamento degli accordi di Bretton Woods, oltre che una significativa opportunità per inserirsi nelle nuove rotte commerciali che si aprono verso l'Oriente. Per l'Italia si tratta inoltre di rafforzare ulteriormente i rapporti economici con la Cina, tenuto conto anche della forte intensificazione del ritmo di crescita degli investimenti cinesi in Italia negli ultimi anni, che interessano ormai interi *asset* strategici e aziende chiave come Terna, Saipem, ENI, ENEL, Telecom Italia e FCA, solo per citarne alcune. Tra gli obiettivi di medio e lungo periodo dell'adesione italiana si possono annoverare le opportunità offerte per l'internazionalizzazione delle imprese italiane e la partecipazione a gare d'appalto per i progetti finanziati dalla Banca. asiatica può costituire un indispensabile volano per attrarre i numerosi Paesi coinvolti dalla nuova via della seta, offrendo loro maggiori prospettive di sviluppo e la possibilità di dotarsi finalmente di capitale fisso in misura assai ingente. In questa prospettiva il nostro Paese si colloca perciò in una posizione di importanza fondamentale. In quanto azionista dell'AIIB, l'Italia parteciperà alle riunioni degli organi di governo della Banca, nei quali sarà rappresentata dal Ministro dell'economia, e potrà disporre di un proprio rappresentante nel *board* dell'Istituzione, avendo dunque la possibilità di prendere parte attiva nei processi decisionali della nuova struttura. Si fa presente che una rapida ratifica della nostra partecipazione alla Banca consentirebbe al nostro Paese di essere rappresentato, con diritto di voto, già alla prima riunione del consiglio d'amministrazione che, come è stato detto La ratifica in tempi brevi consentirebbe poi al nostro Paese di avvalersi dei vantaggi riservati ai soci fondatori, ovvero un'attribuzione di 600 ulteriori voti rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione azionaria in senso stretto, oltre alla possibilità di concorrere alla definizione dei vertici della struttura di *governance*, in particolare del direttore esecutivo e dei vice direttori.

per mettere in discussione quelle vecchie istituzioni finanziarie. Il problema che ci troviamo di fronte è che in questa Banca, nella quale l'Italia è voluta entrare,

quale sia la politica che vuole attuare l'Italia, perché il vero problema è quello. Dove ci vogliamo collocare? Siamo ancora i fedeli alleati atlantici di una volta o vogliamo provare a fare un cambio di passo?

Grazie In questa continua incertezza ci troviamo a dover decidere la partecipazione italiana con circa 2,5 miliardi.

Dove vogliamo collocarci? Non è chiaro. C'è stato qualcuno che in passato riusciva sempre a muoversi in uno strano modo, quando eravamo amici sia degli israeliani che dei palestinesi: ovviamente stiamo parlando

Leggiamo che gli Stati Uniti vogliono aumentare gli stanziamenti per la difesa per contrastare la predominanza che si sta accentuando dell'asse russo‑cinese. E noi ci troviamo ancora una volta in una posizione di limbo. Il vero problema è capire noi chi siamo e dove vogliamo collocarci: questo è il motivo per il quale abbiamo profonde difficoltà a capire bene qual è la posizione dell'Italia. Non riusciamo

in modo chiaro qual è la posizione che l'Italia vuole assumere nello scacchiere geopolitico mondiale per riprendere la sua capacità di essere una Nazione forte. Noi siamo una Nazione straordinaria, ma abbiamo ceduto completamente le armi a qualcuno che teoricamente è sopra di noi, ma non ha la forza, la capacità, l'energia, la voglia di essere come noi. Allora dove siamo?

Grazie Grazie

ciò che doveva essere detto anche per affrontare le questioni sollevate nell'intervento che abbiamo appena ascoltato. Il contesto nel quale noi intendiamo collocarci è quello dello sviluppo della cooperazione internazionale e del massimo sviluppo degli scambi e del commercio in una dimensione globale, in un contesto nel quale il superamento del vecchio mondo è un dato di fatto, ma in larga misura è ancora necessario costruire i soggetti che in una dimensione internazionale debbono gestire il il nuovo mondo, quello che è uscito dal superamento del vecchio. Costruire banche di cooperazione per il credito adeguate alla dimensione internazionale - penso, ad esempio, ai Paesi dell'America latina che hanno già un istituto di questo tipo con la partecipazione del nostro Paese - così come costruire uno strumento come quello che viene proposto adesso per la realtà asiatica è assolutamente essenziale perché l'Italia,

abbia il ruolo di equilibrio che le compete, essendo uno dei principali mercati mondiali e uno dei protagonisti della vita dell'economia globale. Non c'è bisogno di aggiungere altro, se non che

Aderire a questa proposta non ci trasforma in nemici né degli Stati Uniti né del Giappone. Si tratta di uno strumento rispetto al quale quei Paesi hanno espresso una valutazione dei loro interessi nazionali e della prospettiva mondiale diversa da quella che noi coerentemente sosteniamo. Questa è la sostanza. Non credo sia importante sostenere altre ipotesi che non trovano accoglimento in un contesto nel quale - ripeto - non ci sono secondi fini. Questa Banca si costruisce per fare in modo che investimenti infrastrutturali

Signor Presidente, la breve discussione generale e la replica del Governo hanno sollevato spunti interessanti di riflessione dopo la buona relazione

con un'azione e un'attività che valuteremo poi nel tempo, un vuoto in quel nuovo mondo che si è venuto a creare per l'effetto di una globalizzazione che noi italiani non sempre abbiamo compreso in tempo. Infatti, non abbiamo percepito in tempo come quella globalizzazione avrebbe cambiato inevitabilmente il destino della nostra economia. Per volontà della Repubblica popolare cinese, però, l'idea di fondo è proprio quella di colmare l'enorme divario di investimenti nel settore delle infrastrutture e sviluppare una nuova via della seta sulla sulla scia di una antichissima tradizione, anche economica, che ha unito i nostri continenti, per ricollegare l'Asia al Vecchio continente che siamo noi. Ma come si colloca l'Italia in questo ambizioso progetto? Seguendo l'esempio del Regno Unito, siamo stati tra i primi Paesi europei ad aderire al progetto della nuova banca, contemporaneamente a Francia e Germania, aspirando così a essere soci fondatori e soprattutto a far parte della *governance* che è la cosa più importante di questa nuova banca, prendendo anche parte, in veste di Paese membro, alle riunioni del consiglio dei governatori e alla prima riunione annuale della Banca, prevista per i giorni 25 e 26 giugno. Come però spesso accade, pur avendo aderito di concerto lo scorso marzo, Francia e Germania sono stati più solerti di noi nella ratifica e i loro rappresentanti sono già membri di quel *board*, mentre l'Italia ad oggi è rappresentata solo in maniera informale. Speriamo, quindi, che la ratifica di oggi ci aiuti a recuperare questo *gap*. In ogni caso, al di là di rimarcare il *trend* tipicamente italiano di arrivare ultimi anche quando potremmo essere in prima linea, il mio Gruppo, quello dei Conservatori e Riformisti, come opposizione pensa che in questa occasione più che mai il nostro ruolo debba essere quello di stimolare il dibattito su alcune questioni fondamentali. Inutile ricordare che siamo in un momento storico più che delicato. La creazione di questo nuovo istituto avrà inevitabilmente delle ripercussioni estremamente forti sull'economia globale, e si metterà in competizione con il Fondo monetario internazionale - questa lo considero un'ottima notizia con gli indirizzi di Stati Uniti e Giappone, che infatti non hanno aderito e si sono dimostrati sin dall'inizio molto critici. Come il vice ministro Morando, anch'io considero questo un errore, che ripete

La domanda però è la seguente: riusciremo a tenere ben presenti i nostri interessi e a massimizzare i benefici che possiamo e dobbiamo trarre da questa occasione? Riusciremo a proteggere l'eccellenza che è il marchio di fabbrica del *modus operandi* delle imprese italiane, soprattutto delle piccole e medie imprese, per le quali la conquista di una fetta del mercato asiatico costituirebbe un poderosa ventata di ossigeno? E dico questo anche perché, dal lato opposto, il pericolo è un altro: gli investimenti cinesi all'estero sono una realtà in crescita esponenziale. Sono iniziati con il lancio negli scorsi anni di un programma importante per l'internazionalizzazione delle imprese cinesi. Nel 2014, signor Presidente, il volume degli investimenti cinesi all'estero aveva superato per la prima volta quota cento

Solo nei primi cinquanta giorni del 2016, le acquisizioni industriali cinesi all'estero hanno superato il valore di 81 miliardi di è il segno di una grande vitalità. Gli esperti cinesi, infatti, ci spiegano che il programma di internazionalizzazione delle imprese dovrà servire a creare una sorta di piattaforma per aumentare la presenza dei gruppi cinesi nell'economia globale. E noi cosa facciamo? Nella corsa alle fusioni e acquisizioni, la Cina ha un debole per l'Italia, tanto che da sola ha rappresentato il 27 per cento di tutti gli investimenti esteri affluiti nel nostro Paese nel 2014, e non è poca cosa. La lista delle aziende italiane partecipate da colossi cinesi è lunghissima - sono più di 300 - e gli investimenti non si arrestano. Anzi, l'acquisizione di Pirelli da parte di ChemChina, l'hanno scorso, dimostra che il tiro è stato alzato e che la dimensione degli investimenti si è fatta più importante. Tre quarti delle aziende partecipate si trovano nell'Italia

L'investimento più corposo nel nostro Paese è stato quello del gigante energetico cinese State Grid, la maggiore società elettrica al mondo, che nel 2014 ha speso oltre 2 miliardi di euro per rilevare il 35 per cento di Cassa depositi e prestiti Reti,

politica occorra per poter collocare correttamente l'internazionalizzazione delle imprese cinesi anche nel nostro Paese, in maniera tale che sia a favore della nostra economia, e quanto soprattutto resti da fare per accompagnare al meglio le imprese italiane nell'acquisizione di quei mercati così importanti. All'entità degli investimenti cinesi nel nostro Paese si aggiunge la massiccia presenza delle merci cinesi. Non abbiamo compreso in tempo cosa sarebbe Nonostante l'Europa abbia sino ad ora negato alla Cina lo *status* di economia di mercato, è ben possibile che prima o poi questo le venga riconosciuto; il che comporterà l'eliminazione dei dazi che oggi proteggono il Vecchio continente dall'invasione manifatturiera asiatica. Il grande interrogativo quindi rimane: come saprà il nostro Paese farsi valere in un contesto così competitivo? Come potrà sfruttare al massimo l'opportunità di essere membro fondatore di questo organismo che sarà così importante per lo sviluppo economico globale? Come difenderemo la storia economica e le aziende italiane? Con il voto favorevole io mi auguro che non solo questo Governo ma tutte le istituzioni preposte difenderanno le imprese italiane, mandando in quell'organismo

quindi, annunciamo subito il nostro no, spiegandone però le motivazioni. In realtà mi sono chiesta subito perché l'Italia dovrebbe ratificare un accordo che istituisce una banca che è stata già fondata a Pechino e soprattutto perché dovrebbe legittimare una istituzione finanziaria internazionale proposta dalla Repubblica popolare cinese. A detta di alcuni osservatori del settore, la banca in questione dovrebbe contrapporsi al Fondo monetario internazionale, alla Banca mondiale, all'Asian development bank, ovvero quella banca regionale istituita nel 1966 per proporre lo sviluppo delle Nazioni asiatiche e dell'area del Pacifico. Tuttavia, mi pare di avere capito che la Banca asiatica, a parte lavorare in stretto contatto con le citate Asian development bank e Banca mondiale, intenda collaborare anche con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e con la Banca europea per gli investimenti.

forse perché è l'unico libero e scevro dalle logiche dei partiti che ne condizionano perfino i contenuti - quanto segue: «Mentre aumenta il peso degli investimenti cinesi nella Penisola, il Tesoro ha ufficializzato la partecipazione di Roma al capitale della Asian infrastructure investment bank, studiata come alternativa alla Asian development bank e più al sistema di istituzioni internazionali sostenuto dagli Stati Uniti». Personalmente, leggendo queste poche parole, ho capito che qualcosa non sta andando per il verso giusto, o perlomeno non mi convince. Così come non ci convince la nota del Ministero dell'economia, dalla quale si legge che l'Asian infrastructure investment bank (AIIB), quale nuova banca d'investimento che lavorerà con le banche multilaterali di sviluppo e di investimento esistenti, può svolgere un ruolo di rilievo nel finanziamento dell'ampio fabbisogno infrastrutturale dell'Asia. L'obiettivo sarà promuovere lo sviluppo economico e sociale nella regione e contribuire alla crescita mondiale. Ora io mi chiedo qual è il vero motivo che ha spinto Parigi, Berlino e Roma a operare in stretto raccordo con i *partner* europei e internazionali per fondare questa banca. Forse dobbiamo dire, noi del Movimento, che la verità risiede nel fatto - direi non indifferente - che la Repubblica popolare cinese conti partecipazioni rilevanti anche in Saipem, in Assicurazioni Generali, ENI, ENEL, Prysmian, Telecom Italia e Fiat Chrysler Qualcuno ha scritto come sia abbastanza evidente che la decisione italiana non sia indipendente dalla scala crescente che gli interessi economici cinesi stanno assumendo in Italia. Ricordo a tutti che il *manager* cinese, Yunpeng He, è entrato per la prima volta nel consiglio di amministrazione di un'azienda quotata a Piazza Affari; e non mi riferisco soltanto a una società dal forte peso strategico; mi riferisco alla partecipata dello Stato italiano Terna, che - come abbiamo ben scritto - ha in pancia la rete elettrica della nostra Penisola.

siglare certi accordi con la Cina per fare un favore ad alcune società partecipate italiane. Ricordo che il colosso pubblico di Pechino State Grid Corporation of China ha comprato per 2 miliardi di euro il 35 per cento di Cassa depositi e prestiti Reti, controllata di Cassa depositi e prestiti, che detiene a sua volta il 30 per cento di Snam e, appunto, di Terna. Ricordo ancora che molte altre aziende della Repubblica popolare cinese hanno messo a segno in Italia 13 operazioni per un controvalore di 4,9 miliardi. Tra l'altro, vorrei solo riflettere con voi su un aspetto che mi ha colpito, ovvero quello secondo cui l'Asian infrastructure investment bank pare essere stata progettata come un'istituzione tra Governi per lo sviluppo regionale in Asia, che ha il fine principale di offrire sostegno finanziario per la costruzione di infrastrutture nei Paesi in via di sviluppo della regione. Ripeto: sostegno finanziario per la costruzione di infrastrutture. Quindi, stiamo dicendo che l'Italia ha deciso di promuovere - tra l'altro conferendo una quota pari a 2.571.800.000 dollari statunitensi, costituita per l'80 da capitale a chiamata e per il 20 per cento da capitale da versare - lo sviluppo economico finanziario globale e regionale asiatico, attraverso l'investimento in settori come quello dell'energia, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle infrastrutture rurali, dello sviluppo e della logistica urbana. Peccato che queste quote di partecipazione siano in dollari - badate bene - il che lascia ancora milioni di dubbi, e sono state determinate mediante una formula che fa riferimento al prodotto interno lordo. Non credo che l'Italia navighi nell'oro. Eppure, mi risulta che sia il quinto Paese non regionale, dopo Germania, Francia, Brasile e Regno Unito ad avere sostenuto questa iniziativa, iniziativa, che in termini di costi lascia dubbi anche agli esperti del Servizio del bilancio, che hanno fatto le seguenti considerazioni, soprattutto con riferimento alle azioni a chiamata. Così si legge: «Pur considerando che il relativo pagamento ha carattere eventuale, andrebbe chiarito con quali modalità e sulla base di quale possibile tempistica si potrà far fronte a tale impegno nel caso in cui si rendesse necessario il versamento richiesto a seguito della sottoscrizione. Con riferimento - invece - alle risorse utilizzate, disponibili sul conto corrente di Tesoreria 20013, andrebbero acquisiti elementi volti a verificare gli effetti prodotti dalle disposizioni in esame in termini di fabbisogno, in relazione agli utilizzi delle medesime disponibilità, già scontati ai fini delle previsioni tendenziali». Inoltre, si prende atto di quanto indicato dalla relazione tecnica circa la possibilità di far fronte, con le medesime risorse,

potenzialmente è favorevole a un modello alternativo a quello atlantista, nutriamo molti dubbi sull'adesione dell'Italia alla Banca asiatica per gli investimenti. I motivi che ci spingono a nutrire così tanti dubbi sono sostanzialmente i la coscienza e percezione concreta di come il Governo Renzi voglia comunque stare con due piedi in una scarpa (la scarpa si chiama Italia, mentre i lacci si chiamano Cina e USA); la constatazione che la seconda lettura di questo provvedimento non ha suscitato alcun ravvedimento operoso da parte della maggioranza, che non ha nemmeno voluto tenere in considerazione la stranezza della quota partecipativa dell'Italia, che - ricordo ai cittadini - non verrà versata con moneta corrente, ma in dollari, con potenziali effetti negativi per la nostra finanza pubblica nel caso di inasprimento dei tassi di cambio. L'ultimo motivo - ma non per importanza - è dettato da un condizionale utilizzato il giorno 25 maggio dal relatore Pegorer, quando, nell'illustrare il provvedimento in esame, affermava in realtà l'adesione del nostro Paese all'Istituto potrebbe costituire una scelta strategica importante, anche con riferimento al nuovo quadro finanziario globale, segnato dal moltiplicarsi dei soggetti e dal superamento degli accordi di Bretton Woods, oltre che una significativa opportunità per inserirsi nelle nuove rotte commerciali che si aprono verso l'Oriente, sulla cosiddetta nuova via della seta. Bene, proprio perché «potrebbe» costituire una scelta strategica - e quindi non è ancora una scelta sicura il Movimento 5 Stelle non si sente di appoggiare un condizionale, ma preferisce votare no e rimanere con i piedi per terra. Invita, infine, l'Esecutivo a non siglare più accordi volti a curare oggi gli interessi dei cinesi o domani degli americani. Inizi a pensare seriamente e fattivamente agli interessi degli italiani, visto che sono loro i nostri e i vostri datori di lavoro.

È stato giusto anticipare l'approvazione del provvedimento all'inizio di seduta, in modo da poter arrivare in tempo perché l'Italia sia rappresentata alla prossima riunione di questo importante organismo. Noto, però, che - com'è stato evidenziato - se lo si fosse fatto prima, l'Italia

del Parlamento, la cui funzione legislativa viene vista come il principale ostacolo alla velocità e alla tempestività dei provvedimenti - lo sappiamo bene - sta

il Governo è stato fermo otto mesi, dalla firma del protocollo a quando il Governo si è scomodato a presentare il disegno di legge

Le ragioni sono state espresse bene e in modo compiuto nella relazione del collega Pegorer, relatore di questo provvedimento. Devo dire che, al di là di ogni altra cosa, tali ragioni stanno veramente nei titoli sui quali vertono gli articoli e sui quali è chiamato a impegnarsi il nostro Paese all'interno dell'istituzione

Con chi stiamo? Stiamo con l'Europa, perché i più grandi Paesi europei sono qua. Perché abbiamo la quinta quota in questa banca? Perché il nostro è il quinto prodotto interno lordo tra i Paesi che partecipano a questa società. Per quanto possiamo parlare male di questo Paese, fra tutta la compagnia di giro che interviene (e ci sono dei *player* molto forti), il nostro Paese è molto considerato. che condivido le annotazioni un po' critiche del senatore Malan circa la tempistica, che abbiamo già visto diverse volte per altri provvedimenti. Pur tuttavia la tempistica in questo caso non complica particolarmente la situazione, perché la prima riunione del consiglio di amministrazione è prevista per il 25 giugno e, quindi, facciamo in tempo a essere a pieno titolo

riguarda migliaia e migliaia di imprese che operano pressoché in tutto il territorio nazionale, poiché numerose sono le Regioni italiane che hanno coste su cui hanno visto crescere attività. [**Presidenza del vice

Il tema di fondo è se le imprese che operano in queste zone devono, possono proseguire le loro attività, spesso spesso antichissime. Ci sono zone di turismo storico: cito quelle della Versilia, che sono state tra le prime in Italia, nel secolo passato e forse anche prima, a sviluppare attività turistiche che poi man mano si sono estese ad altre parti del Paese. Chi da decenni, alcuni anche da più di cento anni, pratica delle attività, pagando dei canoni, rispondendo a tutta una serie di esigenze e svolgendo anche attività di tutela ambientale

Chiarisco subito che, per quanto riguarda pagamenti e canoni, la discussione può essere aperta. Ci sono casi in cui si paga troppo poco? Probabilmente sì. Del resto, ogni tanto in Italia scopriamo che anche in grandi aree metropolitane patrimoni immobiliari e case in zone di pregio sono a disposizione di persone (importanti o comuni) per pochi euro. È quindi possibile che ci siano anche casi di concessioni o di canoni troppo esigui. Dunque, da questo punto di vista, è giusto che i pagamenti siano commisurati alle potenzialità di ricavo economico.

hanno guadagni ovviamente stagionali, trattandosi di un'attività che non si può svolgere tutto l'anno, come è assolutamente evidente. Ebbene, anche questo settore potrebbe essere sconvolto dalle procedure di gara, che potrebbero vedere anche organizzazioni più ampie. C'è addirittura chi parla di multinazionali appositamente attrezzate per proporre condizioni migliori, forti della loro dimensione, capaci di spalmare oneri, costi o prospettive di guadagno su strutture più ampie e su tempistiche più lunghe.

Abbiamo visto che anche gli altri Gruppi hanno presentato delle mozioni che apparentemente convergono su alcuni obiettivi, ma solo apparentemente.

odierno. Anche la senatrice Granaiola ha partecipato con me e altri colleghi parlamentari a decine di assemblee in tutt'Italia con gli operatori del settore, che rappresentano una risorsa occupazionale, una risorsa d'investimenti, una realtà economica e produttiva. Si dice di puntare sul turismo, sulla cultura e sull'accoglienza della nostra Nazione,

la proprietà del litorale rimane allo Stato e si tratta di regolamentare le attività che avvengono in prossimità del litorale, permettendo allo Stato

Ammesso che vinca il rimanere in Europa e non la Brexit, l'Europa ha dovuto accettare una serie di condizioni

l'Inter e forse anche il Milan, mentre gli americani si sono comprati la Roma (ma non sono americani abbastanza ricchi). Non vorrei che il mio Paese fosse comprato a pezzettini.

non già in tutti i Paesi dell'Europa. Quindi, possiamo e dobbiamo invocare una specificità. Nella nostra mozione - e non scendo nei dettagli - citiamo il fatto che il Portogallo e la Spagna

balneare, con delle concessioni lunghe, e noi no? Perché la Gran Bretagna, per rimanere in Europa, sconta delle condizioni migliorative su temi delicatissimi? Si può stare in Europa e dire che abbiamo delle specificità.

ci stiamo occupando della realtà quotidiana del Paese. È in corso la stagione turistica e anche oggi molta gente ha lavorato in tutte le nostre spiagge. Il Parlamento tuteli con regole chiare, certe e trasparenti, e con oneri adeguati al ricavo di mercato, questo settore produttivo. Sarà anche un modo di rispondere a quell'accusa di distrazione

In questo momento la problematica legata alla direttiva Bolkestein è una di quelle che sta affliggendo maggiormente il settore del turismo e in particolar modo quello balneare,

che ne fa parte. Nel caso dell'Italia, la situazione delle imprese balneari sta rischiando veramente il collasso e rischia davvero di mettere in ginocchio il settore del turismo, di cui tutti noi

Oggi abbiamo la possibilità di dimostrare ai nostri concittadini, a quei 30.000 concittadini che stanno aspettando una risposta dal Governo e da questa Assemblea parlamentare, che intendiamo dare quella risposta e quella speranza, che tutti auspicano di veder realizzata il più velocemente possibile.

la direttiva 2006/123/CE, cosiddetta Direttiva Servizi, ha individuato il regime concorrenziale, come il sistema attraverso cui erogare i servizi e svolgere le attività commerciali e intellettuali, con l'obiettivo di consentire una libera circolazione dei servizi e di garantire la libertà di stabilimento; in particolare, la direttiva contiene disposizioni volte a favorire una competizione trasparente e accessibile ai diversi operatori, anche nel settore delle imprese balneari, che viene considerato assoggettabile a gare e, dunque, a procedure ad evidenza pubblica; la normativa italiana si è dimostrata, da subito, confliggente con le disposizioni comunitarie, ed il legislatore negli ultimi dieci anni ha affrontato il tema attraverso disposizioni transitorie fondate sul principio della proroga, del tutto discutibili dal punto di vista della legittimità, ma soprattutto carenti di una visione di lungo periodo per un settore così strategico per il nostro Paese. In questi anni, per non prendersi la responsabilità di fare delle scelte, è stato creato un regime ambiguo per gli operatori economici, provocando ripetuti conflitti e contenziosi giudiziari in occasione del rinnovo automatico delle concessioni così come di procedure di evidenza pubblica. In più di un'occasione, i tribunali amministrativi, aditi per disciplinare i contenziosi, hanno rilevato nei rinnovi automatici una possibile restrizione ingiustificata alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, non consentendo agli operatori di competere in condizioni di equità, attraverso attraverso procedure di selezione imparziali e trasparenti. In maniera particolare, il riferimento lo facciamo al TAR Sardegna e al TAR Lombardia, che hanno ritenuto i rinnovi automatici molto estesi e potenzialmente colpevoli di sottrarre al mercato beni di notevole rilievo economico. I giudici amministrativi hanno, a loro volta, fatto ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea, sollevando ben due questioni pregiudiziali, per verificare la compatibilità della normativa nazionale riguardante il rinnovo automatico delle concessioni con gli articoli 49, 56 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con i principi, dunque, di libertà di stabilimento, protezione della concorrenza ed eguaglianza di trattamento tra operatori economici, nonché con i principi di proporzionalità e ragionevolezza. alla questione si è già espresso l'Avvocato generale della Corte di giustizia dell'Unione europea, il quale ha formulato le conclusioni generali sul caso proprio alla fine del mese di febbraio 2016. Le conclusioni non costituiscono un atto giuridicamente vincolante. Tuttavia, nella grande maggioranza dei casi trattati, ben 12 costituiscono la base della successiva sentenza della Corte di giustizia. L'Avvocato generale della Corte di giustizia ha confermato i dubbi dei tribunali amministrativi circa la compatibilità dei rinnovi automatici con la normativa comunitaria, la direttiva non consenta tale tipo di operazioni. Lo sfruttamento del demanio pubblico marittimo e lacustre viene infatti ricompreso tra i servizi di cui si occupa direttamente la direttiva: del numero limitato delle autorizzazioni disponibili a causa della limitatezza delle risorse naturali, esso deve essere gestito attraverso procedure di selezione imparziali e trasparenti, con una durata limitata. Si sottolinea come la materia trattata concerna beni e risorse di particolare rilievo rilievo nel nostro Paese, quali le spiagge, i mari e i laghi. Oltre alla necessità di assicurare la concorrenza, come previsto dalla normativa comunitaria, altre considerazioni dovrebbero spingere il Governo ad intervenire per modificare la normativa vigente, al fine di garantire non soltanto la maggiore trasparenza possibile nelle procedure pubbliche di selezione, ma anche la garanzia di una piena accessibilità per tutti i cittadini al demanio pubblico marittimo e lacustre e la tutela dell'ambiente Al tempo stesso, è necessario prevedere che le modalità di assegnazione dei beni demaniali non comportino rischi per i lavoratori impegnati nel settore, ma anzi rappresentino nuove opportunità di crescita di posti di lavoro, che siano presenti dei limiti stringenti al numero di concessioni assegnabili ad un stesso soggetto e che si definiscano opportune forme di indennizzo per gli investimenti realizzati e si tenga conto delle professionalità acquisite. Per questi motivi chiediamo al Governo di impegnarsi, con interventi normativi, al fine di modificare la normativa nazionale in modo da evitare una nuova, ennesima, procedura di infrazione per il nostro Paese, e di attivarsi affinché nelle vengano introdotti criteri in grado di garantire la piena accessibilità da parte dei cittadini al demanio pubblico marittimo e lacustre, la tutela dell'ambiente e del mare, risorse di eccezionale importanza per il nostro Paese, e la tutela dei livelli occupazionali.

Grazie

Grazie Grazie

produzione normativa, come ho detto, da un lato emergenziale e dall'altro sicuramente farraginosa, non ha creato certezze nei confronti degli operatori balneari ed ha lasciato una situazione

ulteriori incertezze nei vari passaggi e nell'esercizio delle varie deleghe da parte di Regioni e Comuni. A fronte di questo quadro normativo abbastanza complicato, dobbiamo innanzitutto metterci nei panni degli imprenditori balneari,

con attività complementari ed accessorie a quelle turistiche, ricettive ed alberghiere, che sono, come si diceva prima, importantissime in tutti i Paesi europei del bacino del Mediterraneo. Tali attività non possono essere abbandonate a se stesse. È un po' come se, nell'ipotesi di dover attuare altri principi normativi, magari discendenti anch'essi dall'Unione europea, a un certo punto si decidesse di chiudere tutte le attività di ristorazione, o comunque di dire a chi opera nel settore del turismo che non ci sono più certezze rispetto a tempi e modalità di esercizio della propria impresa. Nella nostra mozione diciamo non solo che bisogna arrivare ad attuare la delega nel migliore dei modi

Segnalo in particolare che, nei confronti degli operatori che dovessero subire la revoca delle concessioni demaniali, un altro dei principi non attuati a tutt'oggi è quello dell'equo indennizzo.

quali risorse hanno i Comuni per gestire la parte di demanio marittimo non concesso, e per gestire la salvaguardia, la pulizia e la tutela di quei tratti di costa che non sono oggetto di concessioni demaniali. Con quali risorse i Comuni possono far fronte a tutto questo se poi il gettito di quelle concessioni demaniali va allo Stato, e alle Regioni e ai Comuni non viene garantita neanche una piccola parte del gettito di queste concessioni demaniali?

che potrebbero far arrivare sui nostri territori costieri grandi gruppi imprenditoriali che sicuramente possono avere una forza economica maggiore e vanificare la tradizione di queste imprese che hanno scommesso i destini delle proprie famiglie

con il primo provvedimento utile, il rinnovo di quella delega legislativa non esercitata e discendente dall'articolo 11 della legge n. 217 del

durante tutti questi anni (quasi dieci) ha tolto il sonno e la fantasia a più di 30.000 aziende, quelle del settore balneare, che costituiscono una realtà fondamentale per il sistema turistico nazionale, e per due legislature a quei parlamentari che, vivendo sul litorale, hanno dovuto quasi

la proroga al 31 dicembre 2020, messa in discussione da due ricorsi parere dell'Avvocato generale della Corte, hanno gettato nel totale sconforto i nostri concessionari, con una stagione estiva che oltretutto stenta a decollare dati i cambiamenti climatici e i disastri che le varie intemperie hanno causato lungo le nostre coste. Insomma, dopo dieci anni siamo di nuovo al punto di partenza. Non è stata fatta in Europa da parte di tutte le forze politiche quell'azione forte e decisa, non si sono trovate le necessarie alleanze di cui c'era bisogno per far capire che l'incriminato articolo 12 della direttiva, secondo il quale qualora il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato a causa della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, le autorità competenti sono tenute ad applicare una procedura di selezione che garantisca la parità di trattamento dei candidati potenziali. Quindi, l'articolo 12 non può riguardare le nostre concessioni demaniali e i motivi sono soprattutto questi: si tratta di concessioni di beni e non di autorizzazioni che condizionano l'accesso alle attività il bene non è limitato, dato che su circa 8.000 chilometri di coste, solo 2.500 chilometri sono assegnati in concessione. Altri Paesi dell'Unione europea, in particolare la Spagna e il Portogallo, hanno approvato provvedimenti che non tengono conto della direttiva e nonostante ciò non hanno subito procedure di infrazione. Il cammino iniziato in Europa da questo Governo ha bisogno dunque di un forte sostegno di tutto il Parlamento e di uno slancio che faccia valere la specificità del caso italiano e la sua unicità a livello europeo. Soprattutto non dobbiamo aspettare inerti la decisione della Corte di giustizia. Sarebbe un atteggiamento rinunciatario che sicuramente non aiuterebbe ad arrivare ad una definizione positiva della causa. Per questo motivo abbiamo deciso di presentare questa mozione che ripercorre la storia della vicenda, storia ormai nota a tutti. Voglio ricordare che anche nella precedente legislatura era stata presentata una mozione una mozione analoga, che si basa su alcuni principi fondamentali: l'urgenza di mettere in campo tutte le azioni necessarie affinché la proroga al 2020, stabilita con la legge n. 221 del 2012, sia confermata e quindi la necessità per le concessioni in essere di un periodo transitorio adeguato che consenta innanzi tutto all'Agenzia del demanio di effettuare una ricognizione su tutto il territorio nazionale dei beni demaniali e marittimi disponibili e non ancora utilizzati ai fini turistico-ricreativi.

Mi scusi, ma è importante: un periodo transitorio adeguato, e quindi lungo, consentirebbe all'Agenzia del demanio di fare finalmente una ricognizione su tutto il territorio nazionale dei beni demaniali marittimi disponibili e non ancora utilizzati a fini turistico-ricreativi, altrimenti non si riesce a capire come si faccia a dire che si tratta di risorse limitate se non sappiamo neanche quante siano le concessioni concedibili. consentire ai Comuni costieri e rivieraschi di aggiornare o predisporre i piani di utilizzo degli arenili (i cosiddetti PUA), consentendo di assentire nuove concessioni e quindi di incassare nuovi canoni e imposte regionali inerenti; definire canoni equi e sostenibili per tutte le imprese balneari, eliminando dal calcolo di questi ultimi il coefficiente OMI, anche attraverso l'introduzione di criteri di solidarietà, anche suggeriti dalle associazioni di categoria; consentire al Governo di agire in sede comunitaria, sensibilizzando l'Unione europea sulle peculiarità che caratterizzano le imprese del settore turistico-balneare in Italia e per le quali potrebbero essere individuate soluzioni differenti rispetto a quelle previste dalla direttiva servizi, ottenendo dalla Commissione europea il via libera per l'applicazione

quali fattori di esclusione, del sussistere della libertà di stabilimento in ragione della vastità delle risorse naturali presenti lungo le coste italiane e della conseguente possibilità di rilascio di nuove concessioni; far ripartire gli investimenti e creare occupazione in un comparto fondamentale per

Non possiamo eludere poi la necessità di un riordino complessivo di tutta la materia che tenga conto dei principi comunitari, ma anche della specificità del nostro sistema di balneazione, peraltro molto diversificato su tutto il territorio nazionale, e che tenga conto anche dei provvedimenti adottati in alcune Regioni. A tale proposito mi piace citare la legge regionale n. 31 del 2016 della Regione Toscana, contenente disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, emanata con lo scopo di valorizzare il paesaggio e gli elementi identitari della fascia costiera attraverso la qualificazione dell'offerta turistico - balneare con lo scopo di creare adeguate e omogenee condizioni di sviluppo per le micro, piccole e medie imprese turistico - ricreative operanti in ambito demaniale e marittimo, migliorando la qualità delle strutture e dei servizi per la balneazione, migliorando l'accessibilità al mare e valorizzando l'ambiente delle coste toscane. Tengo a precisare che questa legge è stata condivisa dall'ANCI e da molte altre Regioni. In sostanza, con la mozione presentata si chiede al Governo di utilizzare il periodo rimanente fino alla scadenza del 2020 esprimendo in Europa una forte posizione politica tesa a riaprire una negoziazione, anche attraverso alleanze con altri Paesi che si sono già attivati sulla questione, per tutelare il nostro sistema balneare, difendendo la legittimità della proroga al 2020, in linea con la difesa effettuata dalla stessa Avvocatura dello Stato. Quindi non è una richiesta peregrina: la stessa Avvocatura dello Stato ha difeso questa posizione. Si impegna il Governo a valutare con la Commissione europea le motivazioni del diverso trattamento riservato ad altri

prevedere criteri e modalità di affidamento delle nuove concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, che tengano conto della professionalità acquisita nell'esercizio delle concessioni prevedere, in relazione alle suddette innovazioni, un periodo transitorio adeguato per le concessioni in essere di beni demaniali marittimi. Naturalmente, quando si fa riferimento ad un periodo di tempo adeguato non si intende cinque o tre anni, ma, come minimo, mi sembra che si possa affermare che un periodo stabilisca i criteri per fissare i limiti minimi e massimi di durata delle nuove concessioni e stabilisca per i concessionari requisiti e adempimenti volti a comprovare il rispetto delle norme e delle prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, paesaggistica,

Grazie nonché criteri e modalità per il subingresso nelle ipotesi di vendita o affitto d'azienda; g) individui i criteri e le modalità di assegnazione delle concessioni decadute o revocate; h) individui le modalità per la riscossione e per la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra Comuni, Province e Regioni; i) disciplini, fermo restando l'accesso libero alla battigia, le ipotesi di uso o di utilizzo delle aree demaniali. signor Vice Ministro, con l'auspicio che tutte le mozioni che sono state presentate possano essere approvate perché, sostanzialmente, contengono tutte - dico, assolutamente tutte - l'intento di tutelare il nostro sistema di balneazione attrezzato, che, ripeto, è unico e non ripetuto in nessuna Grazie Signor Presidente, è ovvio che anche per il nostro Gruppo la vicenda degli effetti della cosiddetta direttiva Bolkestein, relativi ai servizi nel mercato interno, sulle concessioni demaniali a fini turistico-balneari, fin dal 2006 ha costituito motivo di forte discussione e anche di preoccupazione degli operatori del settore e rappresenta qualcosa di tuttora irrisolto nel panorama giuridico del nostro Paese. Hanno ragione i colleghi che mi hanno preceduto - dalla senatrice Granaiola al senatore Gasparri - a dire che la questione è nuovamente balzata all'attenzione in seguito alle recenti formulazioni dell'avvocato generale della Corte di giustizia dell'Unione europea, il quale, partendo proprio da due casi concreti italiani, ha affermato che quando le concessioni sono limitate a causa della scarsità delle risorse naturali, la direttiva Bolkestein impedisce ai Paesi membri di prorogare in modo automatico la data di scadenza delle concessioni per lo sfruttamento economico del demanio il legislatore italiano, consapevole che sul nostro demanio insistono le attività economiche di migliaia di operatori, anche piccoli, che non hanno le caratteristiche dei grandi colossi internazionali che operano nel settore turistico, ma che pure hanno fatto nel tempo grossi investimenti per migliorare i servizi, svolgendo anche una funzione di controllo e manutenzione delle nostre coste, ha previsto una proroga al 2020 delle concessioni in essere, non intendendo minimamente violare la direttiva comunitaria, non costituendo questo un meccanismo automatico di rinnovo, ma semplicemente un'estensione fino al 2020 della durata delle concessioni esistenti proprio per evitare il grosso terremoto

di trattativa tra le forze politiche. Non dimentichiamo - mi dispiace doverlo sottolineare - che a quel tempo Presidente della Commissione europea era un italiano che si chiamava Romano Prodi. Quindi, non dobbiamo dimenticarci che ci siamo fatti del male da soli dando ascolto a chi le nostre coste non le conosceva, come questo politico Frits Bolkestein, che tra l'altro, colleghi, partecipa alle riunioni dei potenti del gruppo Bilderberg

ai Paesi che affacciano sul Baltico, sarebbe stato un inferno, ma è la dimostrazione che Bettino Craxi a quel tempo aveva ragione anche nell'applicazione di questa direttiva. Qualcuno potrà obiettare che dal 2006 sono trascorsi dieci anni e che questo lasso di tempo potrebbe essere considerato sufficiente per l'ammortizzazione dei costi sostenuti dai concessionari, ma questo non è sempre vero; anzi, per le nostre coste, per i nostri imprenditori non è vero. Al contrario, il rilascio o il rinnovo delle proprio perché ci si rende conto della loro strategica importanza per il turismo nazionale, negli anni sono stati condizionati alla presentazione di progetti sempre più moderni, sempre più attraenti sotto il profilo estetico, sempre più in sintonia con i canoni della sostenibilità ambientale, la qual cosa ha comportato - e giustamente - investimenti enormi per la cui remunerazione non può bastare certamente un decennio di attività. È necessario pertanto, colleghi e rappresentante del Governo, che l'Unione europea si renda conto di queste circostanze e soprattutto si renda conto che noi non possiamo cooperare alla distruzione di un tessuto piccoloimprenditoriale nazionale, con le inevitabili ripercussioni se i concessionari italiani che hanno già scontato all'origine le procedure di evidenza pubblica, che si sono già messi in concorrenza con altri operatori e che hanno acquisito una grossa esperienza sul campo, non potranno contare su un congruo periodo di proroga che travalichi quel termine del 2020 che pure l'Italia ha già previsto per consentire ai concessionari di rientrare dagli investimenti fatti. Ma vi è di più, colleghi. La nostra responsabilità di legislatori che è tanta - deve guardare con attenzione estrema a quello che potrebbe accadere ai nostri piccoli e medi imprenditori nel momento in cui dovessero con i grandi colossi dell'imprenditoria turistica mondiale. Non è cosa da poco. Noi, come Gruppo, riteniamo di dover esercitare questa capacità di rappresentazione profetica della situazione e attivarci in sede europea perché questi aspetti vengano portati

e soprattutto la Spagna e il Portogallo. Vi ricordo che, quando c'è stata la mediazione per approvare la direttiva Bolkestein, i socialisti francesi non l'hanno votata, perché ritenevano che facesse un danno alla loro imprenditoria e alle loro coste, che sono molto sviluppate anche in Francia. Pertanto - e concludo, signor Presidente - noi siamo favorevoli a tutte quelle mozioni che impegnano il Governo ad attivarsi in in ogni modo perché questo settore importante non venga travolto, perché vengano salvaguardati i livelli occupazionali degli operatori del settore e perché venga sostenuta con l'Unione europea ogni utile interlocuzione per far comprendere

e che abbiamo un sistema che deve transitare in maniera indolore e con i tempi necessari verso la nuova prospettiva indicata dalla direttiva Bolkestein. Se ci vuole un altro decennio, ce lo dobbiamo prendere tutto.

e quindi della necessità di tutelarle. Sono un bene paesaggistico e ambientale di primissimo livello e di grande pregio; pertanto tutelate, perché sono parte integrante della nostra capacità economica in materia di turismo. Questo l'abbiamo fatto ad esempio in Sardegna, introducendo un piano paesaggistico che tutela e valorizza l'assetto costiero. L'abbiamo fatto perché forse in Sardegna esistono alcune tra le più belle coste non solo dell'Italia e dell'Europa, ma del mondo.

la gran parte dei quali sono fruibili. Attraverso la pianificazione paesistica, abbiamo introdotto norme che impongono la definizione dei piani di litorale. Nel fare i piani di litorale, abbiamo preservato gli accessi al mare; abbiamo tutelato parti importanti delle coste ad uso turistico-ricreativo assolutamente libere da ogni tipo di vincolo, ivi compreso quello della concessione demaniale a fini turistico-ricreativi, quindi abbiamo una condizione ottimale, anche dal punto di vista dell'insediamento di piccole e piccolissime aziende - qualche volta microimprese - che gestiscono

ci possa essere in Europa un regime così differenziato per cui alcuni Paesi, come quelli della penisola iberica, sono supertutelati anche nella gestione della loro competenza demaniale e altri Paesi, come il nostro, vanno

in modo produttivo e con i tempi che sono necessari per ammortizzare gli investimenti e organizzare in modo adeguato il servizio turistico-ricreativo, soprattutto sulle coste; questi tempi devono essere messi sistematicamente in discussione, anzi essere oggetto

da sfruttare in Sardegna, perché quelle sarde sono di pregio. Non possono quindi essere estromessi senza colpo ferire i cittadini della Sardegna, che già pagano prezzi ormai insopportabili anche sotto il profilo dei diritti

non può funzionare se i nostri beni paesaggistico-ambientali diventano un ambito di mercato per tedeschi, francesi, ungheresi e così via e invece

sarde che devono agire nell'ambito delle concessioni demaniali turistico-ricreative che riguardano le nostre coste? Vogliamo dire che abbiamo

in ambito comunitario affinché l'Unione europea sia finalmente un'Europa dei cittadini, dei popoli e delle Regioni? Lo vogliamo dire o vogliamo ogni

B, a bassa valenza turistica, che - è bene ricordarlo a tutti i presenti in quest'Aula, ma anche a coloro che sono fuori - pagano oneri concessori pari a 1,3 euro per metro quadro all'anno.

Vi è una totale condivisione di anime e sentimento nei confronti dei *supporter* dei concessionari balneari, che vanno rispettati - questo sì

le gare si spostano gli equilibri e perché, in fin dei conti, tutta questa discussione nasce da una marchetta elettorale. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Evidentemente non avete capito che le elezioni le avete perse, perché siete dei miseri conservatori, siete questa roba qui! qui! Noi proponiamo un ordine del giorno di sano buonsenso - perché questo dobbiamo fare, signor Presidente: dobbiamo rimettere al centro il sano buonsenso - in cui chiediamo che si facciano le gare, che si alzino i canoni di concessione chiediamo anche di tutelare gli interessi precipui dell'Italia, perché l'Italia ha tantissime spiagge e non sarebbe bello pensare di essere colonizzati

Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, le mozioni all'esame dell'Assemblea del Senato sollevano il problema del rinnovo delle concessioni demaniali a fini turistico-ricreativi, che interessano gli stabilimenti balneari, ma anche gli alberghi, i campeggi, i porti turistici e gli ormeggi. Stiamo parlando di un comparto economico importante: per le concessioni di stabilimenti balneari parliamo infatti di circa 30.000 imprese, con 300.000 posti di lavoro diretti. Con l'indotto, costituito da piccole e medie imprese, oggi in crisi perché il settore non investe proprio per il clima di incertezza normativa, ci avviciniamo sicuramente quasi ad un milione di posti di lavoro. Dopo che nel 2006 il Parlamento europeo ha varato la direttiva Bolkestein, nel 2009 la Commissione europea, con la procedura d'infrazione, ha messo in mora l'Italia, rilevando l'incompatibilità tra la Bolkestein e le norme nazionali riguardanti il rinnovo delle concessioni demaniali marittime e lacustri. Senza valutare le conseguenze, per chiudere la procedura di infrazione, con due interventi legislativi l'Italia ha abrogato frettolosamente le basi giuridiche costituenti la certezza dei concessionari demaniali, ovvero il diritto di insistenza, cioè la preferenza per il concessionario uscente, e il rinnovo automatico delle concessioni di sei anni in sei anni. a causa del clima d'incertezza creatosi, i concessionari stanno vivendo il periodo più incerto della loro lunga storia, arrestando gli investimenti a discapito anche di un miglioramento dell'offerta turistica complessiva del nostro Paese e i risultati negativi lo stanno a dimostrare. Sono state anche prorogate le concessioni in scadenza al 2009, con una prima scadenza al 2015, spostata poi al 2020, con l'impegno per il Governo - però rimasto inevaso - di legiferare sul riordino della materia entro l'ottobre del 2014. Ad oggi si susseguono testi ufficiosi, sui quali lavorano vari Ministeri, che, se malauguratamente attuati, determinerebbero la fine del comparto balneare italiano. Gli studi comparativi delle norme dei vari Paesi dell'Unione, effettuati dalla Federazione europea delle imprese balneari, evidenziano procedure e regole diverse. Vediamo, ad esempio, cosa succede in Portogallo e Spagna, che sono oggi i nostri maggiori *competitor* a livello turistico balneare. In Portogallo, ad esempio, nel 2007, nel recepire una direttiva europea, è stata approvata la legge dell'acqua, dove vi è il diritto del concessionario uscente ad essere preferito Il rinnovo prevede la durata delle concessioni esistenti fino a settantacinque anni e, lo sottolineo, nessuna procedura d'infrazione è stata posta in essere sino ad oggi. Nel 1998, dopo una sciagurata politica di urbanizzazione delle coste, il Governo blocca ogni tipo di intervento con la legge delle coste, che va a disciplinare e tutelare l'ambiente costiero iberico, demanializzando (espropriando) tutto ciò che era stato costruito sulla costa, ma concedendo in contropartita ai proprietari, una concessione di trent'anni con scadenza nel 2018. Nel 2012 poi, con l'imminente scadenza delle concessioni, i concessionari, operando una forte azione di *lobby* in ambito UE, hanno ottenuto dalla Commissione l'ok per la stessa legge, prodromico ad una nuova legge delle coste, che prevede una proroga secca da trenta a settantacinque anni delle concessioni in essere, senza procedure di evidenza pubblica imposte invece per l'Italia praticamente nel corso dello stesso periodo temporale.

o in via di perfezionamento, da esercitarsi nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della legge. Da sottolineare come la Corte costituzionale spagnola abbia avallato la costituzionalità della nuova legge iberica del 2013, anche in relazione alla proroga delle concessioni demaniali, ben argomentando che la concessione demaniale è configurata come un titolo di occupazione del demanio pubblico e che perciò si tratta di un affidamento di un bene pubblico e non di un servizio. Dunque, in Portogallo come in Spagna, vi è la precisa volontà del legislatore di proteggere e valorizzare le imprese turistiche della costa, che rappresentano un settore strategico per l'economia iberica e portoghese. Anche per la Spagna nessuna procedura d'infrazione è stata posta in essere dal 2013 ad oggi e non è difficile prevedere che mai sarà aperta, visto che la legge della costa va a tutelare gli interessi di molti investitori tedeschi, inglesi e olandesi. è che è indiscutibile che i concessionari di questi Paesi hanno oggi un palese vantaggio nei confronti di quelli italiani, per via della certezza d'impresa acquisita con una proroga consistente, che consente loro pianificazione, investimenti e miglioramento dell'offerta turistica. Come dimostrato dal legislatore portoghese nel 2007 e da quello spagnolo nel 2013 esistono dunque strumenti tecnico-giuridici per trovare la giusta soluzione, ma senza la volontà politica rimangono impraticabili, provocando pareri contrari di tecnocrati che, senza una guida, si impossessano di questo ruolo. Mai come in questo momento di crisi economica le nostre imprese hanno la necessità di essere tutelate e difese dal Governo, dove vi sono sempre più albergatori falliti che decidono di convertire la propria attività ricettiva a quella molto più comoda e remunerativa dell'accoglienza degli immigrati, la maggior parte clandestini, creando un danno devastante soprattutto alle strutture alberghiere vicine. Deve dunque imporsi il primato della politica, una politica che invece in più di una occasione ha mostrato tutta la sua dirompente portata: dall'indiscusso superamento dei vincoli di bilancio da parte di Nazioni *leader* (come la Francia e la stessa Germania) alla proroga delle concessioni autostradali, approvata dal Governo italiano con lo sblocca Italia, sul presupposto dello svolgimento da parte delle stesse di funzioni pubbliche. anche su questo tema, dimostra ogni giorno di più di essere inadeguata di fronte alle molteplici sfide che avanzano, rispetto al perseguimento degli obiettivi inizialmente prefissi per la costruzione dell'Europa da parte dei Padri fondatori, i cui sogni e ideali sono stati traditi. L'Europa è incapace nella gestione dell'immigrazione, ed antepone all'unione politica il perseguimento di un'unione monetaria che, ogni giorno di più con i suoi corollari di politica economica incentrata sull'austerità e sui tagli al bilancio pubblico, ha fatto precipitare un intero Continente in una recessione che sta impoverendo intere popolazioni e Stati, in una crisi di sviluppo di cui non riusciamo a vedere il fondo. La Brexit e la decisione del Parlamento svizzero di annullare la domanda di adesione all'Unione europea sono un campanello d'allarme da non sottovalutare. Oggi dunque il Governo italiano deve operare delle scelte coraggiose, capaci di difendere il substrato vitale e più sano dell'economia italiana,

Crediamo con convinzione - ed è per questo che il Gruppo Lega Nord e Autonomie ha presentato una sua mozione - che anche le nostre imprese balneari meritino una proroga della concessione e il riconoscimento del valore commerciale dell'azienda,

onorevoli colleghi, com'è noto, nel gennaio 2009, la Commissione europea aprì una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia relativa alla normativa in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, in quanto contrastante con la direttiva Bolkestein. Tale direttiva si inserisce nel tentativo di far crescere competitività e dinamismo in Europa ed evidenzia alcune libertà economiche già presenti nel Trattato di Roma del 1957. In verità, la direttiva Bolkestein non intende disciplinare in maniera particolareggiata l'ampio settore dei servizi, ma lascia agli Stati membri la decisione su come applicare nel modo migliore i principi enunciati. In breve, la direttiva sostiene la libertà di stabilimento per semplificare le domande di quanti si vogliono stabilire in un altro Paese dell'Unione per prestare dei servizi, nonché la libertà di circolazione dei servizi

ancora oggi non è consentita piena libertà di circolazione e completa libertà di stabilimento. Al fine di chiudere la procedura di infrazione, nonché di rispondere all'esigenza degli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile che, conformemente ai principi comunitari, consentisse lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare-ricreativa, superando così i rilievi della Commissione, l'articolo 11 della legge

venne prorogato al 15 ottobre 2014, ma ancora oggi non risulta emanato. È grave che i Governi succedutisi negli ultimi tre anni non abbiano ancora provveduto a a formulare una soluzione legislativa che contemperi le esigenze di circa 30.000 aziende operanti in Italia, che danno corpo e vita al settore turistico balneare che rappresenta una fondamentale leva economica delle zone costiere del Paese. L'Italia è attrattore turistico per lo straordinario rapporto con il mare, per il paesaggio marino di insuperabile bellezza, che si estrinseca particolarmente nel Meridione e nelle isole, ma anche il Settentrione, che affaccia sul Tirreno e sull'Adriatico, risulta di incomparabile fascino. La direttiva Bolkestein coinvolge «i servizi ai consumatori, quali i servizi nel settore del turismo, compresi i servizi ricreativi, i centri sportivi, i parchi di divertimento» e le imprese turistico-balneari esistenti nel nostro territorio. La completa disapplicazione della direttiva

della sentenza della Corte di giustizia europea, alcune Regioni stanno cercando di far conciliare le esigenze degli imprenditori balneari con le indicazioni della direttiva. Apparirebbe plausibile in questo contesto la previsione legislativa di un periodo transitorio adeguato a ridurre gli impatti negativi derivanti da un repentino mutamento della disciplina di settore, così come avvenuto anche in altri Paesi europei. Come affermato dalla VI sezione del Consiglio di Stato, che si è espresso con le sentenze del 2012 e del 2014, la disciplina transitoria appare frutto «di una scelta ragionevole del legislatore nazionale, finalizzata non all'elusione della disposizione ma ad una più efficace attuazione (...) dei principi da essa affermati, nel contempo consentendo agli attuali concessionari anche l'ammortamento degli investimenti». Dall'interpretazione di tale sentenza del Consiglio di Stato si potrebbe escludere l'applicazione della direttiva Bolkestein al settore turistico-balneare e ricreativo poiché il bene demaniale non è di per sé un bene produttivo, ma è l'azienda del concessionario a incorporare il bene pubblico nell'azienda privata. È, dunque, l'azienda del concessionario e non la zona demaniale il sito fisicamente rilevato su cui tale azienda insiste La concessione di beni del demanio marittimo non avviene, infatti, per l'acquisizione di servizi da parte dell'autorità concedente, ma viene semplicemente concesso il bene, cioè il demanio marittimo, per l'erogazione di un servizio privato, di un servizio privato, non pubblico, dato che gli stabilimenti balneari sono considerati imprese turistiche dall'articolo 7 della legge n. 133 del 2001. del 2001. Con la mozione presentata dai Conservatori e Riformisti vorremmo pertanto che tutte le imprese balneari, gli organizzatori e gli erogatori dei servizi turistici sulla battigia e sulle coste tirino un lungo sospiro di sollievo. È importante per le economie turistiche marinare balneari avere avere certezze sul piano degli investimenti già realizzati per spronarle a farne di ulteriori, allo scopo di implementare le economie locali che sommate, com'è noto, formano il PIL nazionale, al cui interno sempre più rilevante è il segmento turistico ai fini dell'incremento dell'occupazione, specialmente di quella giovanile. Illustrando le motivazioni della mozione, il collega Bruni ha spiegato che si vuole salvaguardare lo specifico italiano. Insomma,

dobbiamo guardare l'intero sistema con cui in Italia si danno le concessioni. Le concessioni in Italia vengono date nell'interesse dei concessionari, non nell'interesse dei cittadini:

Debora Serracchiani. E intanto il Ministro dice di non dare concessioni perché sta per essere emesso il regolamento. E che cosa succede? Queste proroghe di sessant'anni non solo ingessano il sistema portuale italiano (e per fortuna a Genova questo non è stato fatto anche per merito del presidente Merlo),

avere un'unica frequenza e ripartirsela e si sarebbe risolto il problema delle frequenze in Italia. Invece no, si è fatto questo perché? Perché bisognava dimezzare ancora più i canoni di concessione a RAI e a Mediaset,

in Italia si dice che «tanto non interesserebbe a nessuno». Ebbene, quando è venuto l'amministratore delegato di Telecom in Commissione gli ho chiesto: è vero che se ci fosse un bando di gara per la banda 700 non sareste interessati? Ha risposto che all'indomani avrebbero partecipato alla gara,

concessorio è il male primario di questo Paese, perché si lavora esclusivamente a vantaggio dei concessionari. Arrivando al discorso delle spiagge, ci sono stabilimenti balneari gestiti benissimo, ma quanti sono gestiti male?

in quel momento doveva pensare che si sarebbe potuti arrivare ad una legislazione diversa. Ci sono ammortamenti da fare? Si prendano i bilanci e si guardi quali sono gli ammortamenti. O sono fittizi, sono a parole?

il momento della scadenza delle concessioni sarebbe anche il momento di ridisegnare effettivamente il sistema, con equilibrio, come peraltro previsto per legge, senza che vengano dati due scogli come percentuale di spiaggia libera, non attrezzati, pericolosi, non assistiti, sporchi e così via. Questa è la situazione che andrebbe affrontata. Certo che alcune realtà vanno difese. Mi piace molto, ad esempio, quanto è stato scritto nella mozione del nostro Gruppo, il Gruppo Misto, cioè che non siano sommabili più di un certo numero di

chi partecipa alla gara deve prendersi l'impegno di fare determinati investimenti e tali investimenti non devono essere parole, ma devono essere garantiti come deve essere garantita l'occupazione. Chi dice che se mettiamo a gara gli stabilimenti balneari non aumenta il numero dei dipendenti? Chi dice che non aumenta, ad esempio, il numero dei mesi nei quali si potrebbero utilizzare le spiagge in posti che possono assolutamente utilizzare gli stabilimenti balneari e le spiagge per periodi anche invernali?

*(PD)*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, l'Assemblea del Senato oggi è chiamata ad esaminare un atto di indirizzo su un tema apparentemente di secondo piano ma in realtà fortemente significativo per l'economia del nostro Paese. Al di là di ciò che in quest'Aula si può raccontare circa le finalità delle concessioni, gli stabilimenti balneari (e questo è un dato di fatto) costituiscono per l'Italia un settore fondamentale, data la conformazione geografica della nostra penisola e data la particolare attitudine al turismo delle nostre località costiere. L'economia di intere aree, soprattutto nel Mezzogiorno, risente fortemente degli introiti del settore turistico-balneare, tanto più se si considera che spesso si tratta di comunità la cui sopravvivenza sociale ed economica si regge solo ed esclusivamente sul turismo balneare, stante lo scarso sviluppo industriale e la debole presenza di altri settori imprenditoriali. Nel turismo marittimo, l'hanno detto altri colleghi prima di me, operano circa 30.000 imprese, molte delle quali hanno un carattere familiare. Si tratta di famiglie ed imprese che si trovano da tempo di fronte ad un bivio. Rischiano di vedere vanificati tutti gli sforzi compiuti negli anni e di perdere gli investimenti di una vita, il tutto per delle responsabilità che non sono in alcun modo imputabili a loro stessi. Siamo perciò ad un momento di svolta per il settore. La disciplina normativa necessita di un generale ripensamento (la legge quadro risale al 1993) alla luce dell'entrata in vigore della nota direttiva Bolkestein che, impedendo il rinnovo automatico delle concessioni, porta di fatto al superamento del cosiddetto diritto di insistenza, che aveva caratterizzato l'ordinamento giuridico italiano. Nel 2009 la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione proprio alla luce delle norme vigenti in materia, contestandone la compatibilità con il diritto dell'Unione europea, in particolare con il principio della libertà di stabilimento. La Commissione ha ritenuto che le norme italiane costituissero una discriminazione per le imprese provenienti da altri Stati membri, che si trovavano nella condizione di essere ostacolate dalla preferenza accordata al concessionario uscente. Nonostante la delega al Governo, contenuta nella legge comunitaria del 2010, per emanare un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime, non c'è stato finora un deciso impegno. È mancata probabilmente finora una volontà politica chiara e netta di intervenire nel settore.

il tema delle concessioni demaniali marittime si trascina ormai da troppi anni e le imprese che operano nel comparto sono soggette ad una profonda incertezza normativa.

perciò ad un momento storico. Abbiamo un compito importante, quello di riuscire a trasformare un vincolo in un'opportunità; dobbiamo arrivare ad un ripensamento generale del quadro normativo di riferimento e dobbiamo in questo momento fare uno sforzo

valorizzazione delle attività imprenditoriali e di riconoscimento e tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale,

la qualità paesaggistica e l'insieme degli elementi identitari delle nostre fasce costiere e dei nostri stabilimenti balneari. Non sono tutti uguali: hanno caratteristiche e peculiarità che li rendono unici

la predisposizione di procedure selettive non può rappresentare una modalità per lasciare gli operatori in "balia delle onde" (e mai paragone fu più consono): è necessario, perciò, approvare una norma transitoria per le concessioni in essere, che tenga conto degli investimenti immobiliari e infrastrutturali già effettuati, del valore commerciale della professionalità acquisita in tutti questi anni e ne garantisca il loro riconoscimento e ristoro al termine della concessione. la strategia del doppio binario possa essere l'unica che permette di attuare le norme europee sulla libertà di stabilimento e consenta, nel contempo, di assegnare le concessioni sulla base di una procedura comparativa, questo senza mettere in ginocchio imprese e famiglie che operano nel settore da anni e che con il loro lavoro contribuiscono, oltre che a garantire la sorveglianza delle coste e la tutela dell'ambiente naturale costiero, a mantenere elevato l'interesse turistico delle molte località che il mondo intero ci invidia. Il momento è quindi di urgenza, e, data l'urgenza, sollecitiamo il Governo a farsi promotore in tutte le sedi, nazionali e sovranazionali, di interventi mirati, efficaci e tempestivi. La stagione estiva è ormai iniziata e il settore balneare necessita di una disciplina normativa che lo regolamenti in modo definitivo e stabile. Occorre restituire alle imprese del settore, già soggette agli umori del sole almeno un minimo di serenità normativa, affinché siano messe nelle condizioni di poter effettuare

porti presto a un impegno del Governo per la definizione - insieme al Parlamento - di un quadro normativo certo per i nostri operatori.

Signor Presidente, prima di dare i pareri sulle mozioni e gli ordini del giorno, vorrei riepilogare alcuni aspetti importanti, che peraltro sono stati affrontati anche negli interventi che mi hanno preceduto. Innanzi tutto, è chiaro che la riorganizzazione dell'intera materia delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, come segnalato anche dai senatori che sono intervenuti, presenta profili di rilevanza comunitaria concernenti le procedure di assegnazione delle stesse, alla luce della direttiva del 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. La normativa interna sulle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo è stata contestata dalla Commissione europea, che ha avviato nei confronti dello Stato la procedura di infrazione n. 2008/4908 in ragione del mancato adeguamento all'articolo 12 della menzionata direttiva. Alla luce dei rilievi di incompatibilità con il dettato comunitario, l'articolo 11, comma 1, lettera *a)* della legge del 15 dicembre 2011, n. 217, ha abrogato la disposizione che prevedeva il rinnovo automatico delle concessioni in scadenza e ha inoltre delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime. In conseguenza di detto intervento legislativo, la menzionata procedura di infrazione è stata chiusa il 27 febbraio 2012. Per completezza, giova anche segnalare che il termine di 15 mesi per l'emanazione della legislazione delegata è stato ripetutamente prorogato. Da ultimo, l'articolo 34-*duodecies* del decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge n. 221 del 2012, ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 e in scadenza entro il 31 dicembre 2015. Questo per quanto attiene alla ricostruzione del quadro normativo di riferimento. Detto ciò, deve precisarsi che il ministro Costa ha recentemente evidenziato come sono in corso di definizione le linee guida recanti i criteri per l'emanazione di una legge delega per il riordino generale del demanio marittimo, che sono il frutto di un approfondito confronto e di una serrata trattativa con la Commissione europea, e che si sono sviluppati a seguito della cosiddetta direttiva Bolkestein, per evitare il perpetrarsi di disallineamenti giuridico-legislativi che possono sfociare in ulteriori procedure di infrazione. I lavori interni si stanno svolgendo nell'ambito di un tavolo tecnico-politico, in sede di Conferenza Stato-Regioni, al quale partecipano tutte le amministrazioni cointeressate, aperto ai contributi degli enti territoriali locali, sentendo anche i rappresentanti delle associazioni di categoria dei concessionari. Nel dettaglio, i punti principali per ora richiamati nelle linee guida sono quelli che andiamo qui di seguito a riepilogare e che, a mio avviso, collimano con molte delle osservazioni che qui sono state poste e trasfuse nelle mozioni. In primo luogo, sul tema dei criteri e delle modalità di affidamento delle concessioni, essi sono strettamente collegati all'interesse pubblico, alla valorizzazione delle attività imprenditoriali e al riconoscimento e alla tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, assicurando imparzialità e trasparenza, nonché qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale. In queste linee guida si terrà altresì conto della professionalità acquisita nell'esercizio delle concessioni per finalità turistico-ricreative. In secondo luogo, sarà garantita la pluralità e la differenziazione dell'offerta negli ambiti territoriali di riferimento. In terzo luogo, è prevista la fissazione di un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino, anche in relazione alle innovazioni da introdurre, ivi compreso un ristoro, nel caso di subentro, inversamente proporzionale alla durata del periodo transitorio. Sono tutti temi che sono stati sollevati nel corso del dibattito. Si sta infine valutando la revisione dei canoni concessori, con l'applicazione di valori tabellari a stima diretta secondo la peculiarità dei titoli concessori, che consentano di superare in particolare in particolare le criticità correlate all'individuazione delle opere di facile o difficile rimozione e all'applicazione dei valori OMI ai cosiddetti concessionari pertinenziali. Anche questo è un punto che è stato sollevato nel corso del dibattito. Si tratta del resto, come è noto, delle pertinenze demaniali, cioè di quelle costruzioni realizzate nel tempo da privati in aree di concessione, che risultano incamerate dallo Stato alla scadenza naturale delle relative concessioni, per le quali quindi è stato previsto si pagasse, dalla data del rinnovo delle concessioni medesime, uno specifico canone, fissandolo inizialmente al 300 per cento delle misure unitarie per il relativo calcolo. La legge n. 296 del 27 dicembre 2006 ha previsto che l'Agenzia del demanio rideterminasse il canone annuo relativo alle concessioni che ospitano tali strutture, introducendo un sistema di calcolo commisurato ai valori di mercato. Così si è prodotto di fatto, come evidenziato anche dalla stessa Agenzia del demanio, un notevolissimo incremento dei canoni, non correlabile al contesto delle altre concessioni demaniali marittime, provocando situazioni di insolvenza difficilmente sanabili. Tutto ciò premesso, per quanto riguarda innanzitutto le mozioni presentate, relativamente alla mozione n. 539 a prima firma del senatore Gasparri, il Governo propone, sul primo impegno, la seguente riformulazione: «a verificare con la Commissione europea le implicazioni delle specificità del regime delle concessioni demaniali marittime in Italia, in rapporto con quanto avviene negli altri Paesi europei». Relativamente al secondo impegno, il Governo propone la seguente riformulazione: «a prevedere un adeguato periodo transitorio che accompagni le concessioni demaniali marittime turistico-ricreative in essere verso la piena applicazione della nuova disciplina, ai fini della tutela delle proprie aziende e delle relative ricadute occupazionali, economiche, sociali e culturali». Quanto al terzo e al quarto impegno, il Governo li accoglie nella formulazione proposta. Con queste riformulazioni, il parere è favorevole alla mozione n. 539; altrimenti, il parere è contrario.

prevedere un adeguato periodo transitorio che accompagni le concessioni demaniali marittime turistico-ricreative in essere verso la piena applicazione della nuova disciplina, ai fini della tutela delle proprie aziende e delle relative ricadute occupazionali, economiche, sociali e culturali».

sul primo impegno il parere è favorevole. Sul secondo impegno si propone la seguente riformulazione: «a verificare con la Commissione europea le implicazioni delle specificità del regime delle concessioni demaniali marittime in Italia, in rapporto con quanto avviene negli altri Paesi europei».

mozione n. 595 a prima firma del senatore Barani, sul primo impegno il Governo propone la seguente riformulazione: «a continuare a perseguire un percorso di negoziazione con l'Unione europea con l'Unione europea, per verificare l'applicabilità al tema delle concessioni demaniali balneari del criterio del "doppio binario" (distinguere cioè le concessioni attualmente in vigore dalle nuove concessioni), onde

«a verificare con la Commissione europea le implicazioni delle specificità del regime delle concessioni demaniali marittime in Italia, in rapporto con quanto avviene negli altri Paesi europei».

la seguente riformulazione: «a riferire al Senato su tutte le iniziative che intenda assumere per sostenere in sede europea le legittime istanze degli operatori dei settori citati». Sul punto 2) il parere è favorevole nella formulazione proposta; sul punto 3) si propone di modificare la locuzione:

circa 5.500 ettari a causa di incendi: 3.748 ettari di bosco e 1.878 ettari di macchia mediterranea. Dopo quello che è successo a Pantelleria, devastata dai fuochi, si è creato un momento di grande difficoltà nell'isola:

Ha annunciato che acquisterà droni, autobotti e tutto quello che serve per spegnere gli incendi;

Siamo all'inizio dell'estate e già si sono verificati due incendi molto gravi, come ho detto in premessa.

autobotti che non funzionano e mezzi di qualsiasi tipo, ormai datati, che non sono assolutamente sufficienti per poter

passi immediatamente al Corpo forestale dello Stato per poter meglio coordinare. Basta, quindi, con i Corpi regionali. Parlo della Sicilia. Forse ci saranno Regioni molto virtuose da questo punto di vista,

È da qui che dobbiamo partire per organizzare l'emergenza di domani mattina. Altro che droni e autobotti. Fra cinque anni forse non ci sarà più un albero in Sicilia. Rimarranno solo i forestali stagionali, signor perché adesso ce n'è uno per ogni albero - faccio un'autocritica, che ritengo molto opportuna - e quando non ci saranno gli alberi, rimarranno solo i forestali. bisogna incidere. Occorre poi organizzare un controllo perpetuo del sistema forestale, anche con i servizi segreti, perché si è devastata e distrutta la Sicilia.

darsi che ci siano attività collaterali di chi fa questo mestiere, ma spetta alla magistratura fare questo lavoro, che deve essere accompagnato da una ristrutturazione profonda del Corpo forestale regionale.

Grazie